Presidente, prima di affrontare il merito degli emendamenti e i voti ad essi relativi, ho necessità di

le conseguenze, che vi sono o non vi sono, in dipendenza del voto. Rappresento alla Presidenza che l'emendamento 1.27 concerne una modifica dell'articolo 9

di chiarirci, con riferimento all'emendamento 1.305,

In ordine a queste ripetute richieste di precisazioni al Governo, ad oggi non abbiamo avuto risposta, essendosi detto da parte dell'Esecutivo che questo eventuale chiarimento arriverà quando si affronterà l'emendamento 1.305. Ebbene, signor Presidente, credo non sia di poco conto

sensibile a determinate pressioni politiche, lo abbiamo visto estremamente favorevole verso emendamenti presentati da una componente della maggioranza.

Signor Presidente, già in Commissione ci siamo confrontati su

1.27 e 1.300 che stava affrontando l'onorevole Lucidi riguarda la preclusione, su cui la Presidenza si è già pronunciata. A noi interessa sapere, all'emendamento 1.305 del Governo, quali sono i luoghi destinati per legge alla permanenza temporanea.

rispondere, perché questo non è un punto di poco conto. Il Governo ha depositato, tra gli altri, anche questo emendamento, questo emendamento, l'1.305, che prende in considerazione i centri di permanenza temporanea. In base all'attuale sistema, confermato anche dal decreto‑legge nella sua versione originaria, se un comunitario non si fa identificare ed è necessario procedere al suo allontanamento immediato, è indispensabile identificarlo. La sua identificazione richiede delle strutture di sicurezza che impediscano che si dilegui sul territorio nazionale, in analogia a ciò che avviene con gli extracomunitari e con il sistema previsto dal Testo unico sull'immigrazione. Questo emendamento non riesce a far capire qual è l'obiettivo che si vuole raggiungere. Da ciò la richiesta di chiarimenti al Governo, che noi chiediamo vengano forniti subito, perché si inserisce in un contesto dal quale dipende anche la valutazione degli altri emendamenti. Il quesito è il seguente. Nel momento in cui si dice si dice che «il questore può disporre il trattenimento in strutture già destinate per legge alla permanenza temporanea», se con tale dizione si fa riferimento ai centri di permanenza temporanea l'emendamento è assolutamente inutile, non non sposta e non aggiunge nulla e quindi significa che i CPT vengono confermati anche per le ipotesi di allontanamento immediato dei comunitari.

presentati da colleghi della parte più a sinistra dello schieramento di centro-sinistra sono in qualche modo superati dall'1.305. Ciò farebbe intendere che non si fa riferimento ai centri di permanenza temporanea. Noi allora vogliamo capire quali sono le strutture di trattenimento dei comunitari che non si fanno identificare.

con ciò di cui ci stiamo interessando. Sono, come aleggiato a margine della discussione, quelle che una volta erano le carceri mandamentali? Anche queste non c'entrano nulla, perché sono strutture di detenzione e l'espiazione della pena è una questione totalmente diversa dalla prevenzione di sicurezza a cui sono finalizzati i CPT. Il Governo non può nascondersi dietro un dito, non può nascondersi di fronte ai nostri quesiti, ma anche di fronte alla legittima richiesta dei presentatori degli emendamenti che precedono l'emendamento 1.305 di capire che fine fanno i CPT. Non vogliamo essere presi in giro noi, ma credo non sia giusto neanche che sia preso in giro chi fino a questo momento ha condotto una battaglia contro i CPT che noi non condividiamo, ma che rischia di essere coperta totalmente da una formula che non significa assolutamente nulla prima che il Governo chiarisca qual è l'obiettivo che intende raggiungere.

Si è parlato a lungo di residenza, come se non esistesse in Italia

marzo 1978, n. 59, che obbliga chiunque ospita un cittadino, anche straniero, a denunciare entro 48 ore che risiede presso di lui. Così come l'obbligo di residenza sussiste anche per il cittadino straniero, perché la legge stabilisce che chiunque dimora abitualmente in un determinato Comune ha l'obbligo di comunicare al Comune che vi risiede. Se qualcuno poi affitta un appartamento ad una persona straniera ha l'obbligo, per la citata legge del 1978, di comunicarlo entro 48 ore. Ma quello che più mi ha meravigliato, signor Presidente, è che si siano equiparati, anche negli ordini del giorno, i cittadini extracomunitari ai cittadini europei, dimenticando (e questa è una cosa molto grave) che l'Italia è stato uno dei promotori della Comunità Europea.

il Sottosegretario per l'interno in ordine ad alcuni emendamenti che sono stati proposti anche dalla maggioranza. Allora, è bene sapere

il che sarebbe ancora più grave perché sarebbe una manifestazione abbastanza evidente, addirittura, di selezione e di distinzione razziale. Si tratta,

se andiamo all'estero, perché ci potremmo aspettare uno stesso trattamento dagli altri Paesi della Comunità se dovessimo andare all'estero. Abbiamo predisposto un decreto-legge in cui

Centri di permanenza temporanea, come se i centri di permanenza temporanea non privassero le persone della libertà personale: ciò mi pare abbastanza grave,

dell'opposizione si sia ritenuto che la criminalità in Italia dipenda principalmente dall'allargamento dell'Unione Europea.

Si è dimenticato, inoltre, che proprio questo Parlamento, e proprio per il voto determinante di chi ha lamentato e lamenta oggi in questa sede che la criminalità è dovuta solo all'immigrazione europea

Di tutto questo non si è parlato; si parla di sicurezza e non si dice che in Italia le condanne inferiori a tre anni non vengono praticamente scontate, perché la legge Saraceni prevede che

quando sia possibile applicare una misura di prevenzione personale,

se tale questione debba essere votata, come da noi richiesto, prima di qualunque altro emendamento. Poi il Governo ci dica (se lo vuol dire), non ci dica (se non lo vuol dire), ma dobbiamo sapere, prima di votare qualunque cosa, se queste persone sono o no trattenibili in qualche posto chiamato CPT.

avanzato dai colleghi e che naturalmente deve essere fornita dall'Esecutivo, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo su una norma Sulla base del decreto-legge che stiamo discutendo, ai provvedimenti di allontanamento, per motivi imperativi di pubblica sicurezza (quelli che sono immediatamente eseguiti dal questore), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del Testo unico in materia di immigrazione. Mi riferisco, quindi, ad una normativa che è stata da voi confermata nella scorsa legislatura dalla cosiddetta legge Bossi-Fini. Ebbene, secondo il citato comma 5-*bis*, il questore comunica entro 48 ore al giudice l'adozione del provvedimento. Si svolge l'udienza e il giudice decide entro 48 ore per la convalida. Contro la convalida si potrà poi ricorrere in Cassazione, ma il ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento. A questo punto, vi è una previsione normativa contenuta nel settimo periodo del comma 5-*bis*, che «in attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso» (questo naturalmente si applica anche ai casi che vengono ora considerati nel decreto-legge) decreto-legge) «è trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili». Questa norma, quindi, ipotizza due tipi - se mi consentite di dirlo - di messa sotto controllo dello straniero nei confronti del quale pende un provvedimento di espulsione. La prima messa sotto controllo avviene attraverso il trattenimento presso un Centro di permanenza temporanea, se il termine è così breve per il procedimento di convalida già le norme attuali prevedono che non si ricorra al trattenimento presso un Centro di permanenza temporanea, ma che la persona venga temporaneamente messa sotto controllo con altri mezzi e in altre sedi. Queste sedi mi sembra che non possano che essere le camere di sicurezza dei commissariati. Ma ciò è già possibile sulla base della normativa vigente, che voi avete confermato, che prevede (ove il termine sia breve: qui si parla di 48 ore più 48) un trattenimento diverso da quello presso i classici Centri di permanenza temporanea. La stessa cosa, sulla base dell'emendamento presentato dal Governo, può riferirsi anche al caso di un provvedimento di espulsione che penda nei confronti di persona sottoposta ad un procedimento penale. Qui il termine per la convalida diventa di 15 giorni ed è quindi per questi 15 giorni che si può prevedere il trattenimento presso un Centro di permanenza temporanea oppure, sulla base dell'emendamento presentato dal Governo, un'altra forma di trattenimento che assomiglia a quella già in uso per il termine di 48 ore più 48. La domanda che dobbiamo porci è la seguente: questa forma di trattenimento è rispettosa del criterio di proporzionalità, fissato anche dalla giurisprudenza costituzionale, tra esigenze di sicurezza

per gli stranieri non comunitari si arriva ad un trattenimento fino a 60 giorni. Qui il trattenimento ha un limite molto più basso e può essere svolto, in base a quanto dicevo e in coerenza con la normativa previgente, in due modi:

rispetto a questo problema. Sono stati presentati emendamenti da parte dei colleghi della sinistra che avrebbero messo in discussione i Centri di permanenza temporanea rispetto al problema dei comunitari

che è sfociato nella presentazione dell'emendamento 1.305. Mi auguro che il Governo sia in grado di fornire i necessari chiarimenti. Diversamente, credo che rispetto ad un problema di tale dimensione

Se queste strutture debbano esistere o meno credo debba essere confermato in questa sede con estrema chiarezza da parte del Governo, che dovrà anche chiarire

l'interno*. Signor Presidente, la ragione per cui ritenevo di non dover affrontare tale questione è che nell'ordine dei nostri lavori è molto posticipata rispetto alla discussione

una considerazione rivolta all'intervento del senatore D'Ambrosio, che intendeva interloquire con il Governo che qui rappresento. Al senatore D'Ambrosio che il Governo si è mosso costantemente, con riferimento sia alla stesura del decreto-legge che alla sua trattazione in questo ramo del Parlamento,

perché ciò diventerebbe discriminatorio per i comunitari nonché una sanzione non proporzionata, così come la direttiva vieta L'Italia entrerebbe immediatamente in procedura di infrazione se l'iscrizione anagrafica e la dichiarazione di presenza venissero considerate motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica.

Come i senatori ben sanno, all'interno del comma 3 dell'articolo 13 del Testo unico sull'immigrazione previsto che, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore possa adottare la misura del trattenimento presso un Centro di permanenza temporanea. Questa disposizione esiste

La valutazione da parte del questore in riferimento al luogo in cui trattenere la persona può essere determinata in relazione alla variabilità del tempo del trattenimento. Per tale motivo, abbiamo previsto che, insieme al Centro di permanenza temporanea, citato nell'articolo 13,

Ebbene, senatore D'Ambrosio, se lei lo chiede al figlio delle persone trucidate a Gorgo al Monticano, al marito della signora Reggiani, o a tutti coloro che nel Nord Italia hanno subito rapine in villa, probabilmente costoro le spiegheranno

previste per legge, che invece il Governo, che ha presentato l'emendamento, dovrebbe conoscere

Sono una misura di trattenimento o una struttura alberghiera? Non si può prendere in giro la gente, sopprimendo con un emendamento i centri di prima accoglienza, di trattenimento. Credo che tale misura non possa essere

si possa essere discordanti sul merito di ciò che si propone, però non si possa difettare di chiarezza. Stiamo qui discutendo di limitazioni della libertà personale; allora, se discutiamo di questo, il Governo che presenta un emendamento che si muove su questo piano ha il dovere di scrivere nella legge che propone al Parlamento quali sono i luoghi nei quali si limita, sia pure in forma attenuata rispetto al carcere, la libertà personale. Non è materia da demandare alla circolare di un prefetto o di un capo dipartimento. La Sottosegretario ha detto, di passaggio, e la ringrazio, che entrano in considerazione le camere di sicurezza delle questure: è un passo ulteriore. Registro che una struttura, che è dedicata al fermo amministrativo di polizia

rettificando questo emendamento in modo chiaro, quali sono le strutture; in materia di libertà personale non ci si può affidare a nulla se non alla legge dello Stato.

e chiedo a lei di esercitare la sua facoltà di proporre all'Aula la questione sospensiva, perché mi pare che l'elemento nuovo ci sia - eccome - per giustificare la richiesta: le dichiarazioni reticenti

Signor Presidente, è evidente che il Presidente dell'Assemblea raccoglie il senso

possa essere in grado di dire, non solo ad una parte o all'altra, al vice presidente Calderoli o al presidente Castelli, ma all'Assemblea e quindi anche a lei, ciò è opportuno o meno. Infatti, se effettivamente vi fosse un'opportunità oggettiva per migliorare il testo, allora anche noi potremmo essere d'accordo, ma se questa opportunità non c'è, se non vi sono le condizioni, se non serve ed è una perdita di tempo, allora, anche noi riteniamo sia del tutto inutile. Però, nessuno più del presidente Bianco può esprimere all'Aula un'opinione, non solo autorevole, ma anche valida.

La seduta è sospesa.

Nel corso dei lavori alcuni colleghi hanno sollevato questioni interpretative che erano state già poste in Aula. Il Governo, da parte sua, ha fatto presente

per acquisire le valutazioni di tutti i Gruppi sull'argomento di cui stiamo discutendo e sulle questioni connesse. Pertanto, signor Presidente, se così fosse, se tale esigenza fosse mantenuta e confermata, come mi sembra, dal Governo,

Signor Presidente, credo che la sospensione che abbiamo ottenuto sia stata estremamente utile per fare chiarezza. le spiegazioni che ci sono state date dovessero essere formalizzate nei termini in cui ci è stato detto da parte del Presidente e del Governo, noi saremmo pronti anche a sostenere l'emendamento, purché, ripeto, vi sia specificato quello che ci è stato detto.

sicuramente la votazione di quell'emendamento sarà nel pomeriggio e quindi, nell'intervallo del pranzo, il Governo potrà attivarsi per i contatti con tutte le forze politiche.

e potrebbe rilevare, da questo emendamento fumoso e dalle doppie o triple letture, che invece di garantire maggiore sicurezza si fa maggiore buonismo e maggiore razzismo.

1a Commissione permanente non è riuscita a completare i suoi lavori e si è presentata in Aula senza relatore, il che vuol dire che non c'è stato un adeguato approfondimento. È stata sollevata però una questione delicata e rilevante e rientra nell'ordinaria prassi parlamentare che in questo caso, come ha giustamente chiesto il presidente Bianco, ci sia una breve sospensione, in modo che la Commissione possa approfondire tale complessa questione che presenta più di un risvolto e più di un aspetto.

lo ribadisco - che il Governo, autore di questo emendamento, lo riscriva, facendo capire qual è la formulazione definitiva. Peraltro, se effettivamente la formulazione definitiva fosse quella anticipata dal sottosegretario Lucidi, credo si porrebbe inevitabilmente un problema di copertura finanziaria.

sulle espulsioni degli extracomunitari. L'introduzione di questo meccanismo è però al di fuori di qualsiasi copertura possibile e quindi deve essere munito di adeguata copertura, perché le celle di sicurezza dei presidi di Polizia sono assolutamente inadeguate rispetto alle esigenze che questo emendamento intende affrontare.

Presidente, in merito alla questione che è stata sollevata vorrei porre alla sua attenzione anche un profilo regolamentare. La 1a Commissione ha concluso i suoi lavori senza relatore: riunire ora la Commissione,

che il presidente Bianco ha indicato: mi sembra che ciò possa permettere un lavoro più approfondito e un confronto più serrato. Sono d'accordo anche con le motivazioni che il presidente Salvi esponeva poco fa, per cui anche noi siamo favorevoli ad accettare un passaggio in Commissione che ci sembra il completamento di un confronto che non si è potuto effettuare nei giorni scorsi. Presidente, intervengo per esprimere anch'io il consenso sulla proposta avanzata dal presidente Bianco. troviamo in una situazione assai delicata e credo che la sospensione dei lavori, per consentire un confronto ulteriore tra tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione in Commissione, sia assolutamente utile se non si vuole correre il rischio di fare una di quelle frittate per cui poi ci troviamo, addirittura, senza nessun provvedimento.

in presenza di paradossi francamente inaccettabili. *In primis*, il Governo presenta un emendamento che, evidentemente, non è in grado di chiarire. L'aspetto più grave, signor Presidente, è che il legislatore si è sempre sforzato (spessissimo non riuscendovi) di costruire leggi chiare ed inequivocabili.

un emendamento appositamente fumoso, che metterà in difficoltà chi dovrà applicare la legge, per superare problemi di natura politica.

su temi fondamentali della vita del Paese. Abbiamo una sola fortuna: esistono sindaci che da soli, sfidando anche le ire della magistratura di sinistra (la stessa che poi manda a casa i magistrati che osano

Egli deve addirittura sfidare le ire della magistratura, che vuole impedire al sindaco di difendere i propri cittadini! Grazie, signor sindaco!

Presidente, alcune strumentalizzazioni alle quali abbiamo assistito sono assolutamente inaccettabili.

perché legiferare su una materia così delicata, con un decreto, è abbastanza opinabile quando si interviene a caldo e quando ci sono dei fattori esterni che comunque condizionano l'operato del legislatore.

non si è voluto fare prima, inevitabilmente ritorna in un momento come questo. Momento che condiziona i nostri lavori perché purtroppo abbiamo (e lo verifichiamo) degli atteggiamenti preconcetti che invece, in materie sensibili come quelle al nostro cospetto, non dovrebbero assolutamente avere diritto di cittadinanza, perché quando parliamo della libertà, di provvedimenti che incidono sui cittadini comunitari, che sono l'interfaccia di quello che noi rappresentiamo negli altri Paesi dell'Unione europea, dovremmo riuscire a ragionare senza preconcetti ideologici, cosa che invece l'Assemblea ha dimostrato di non riuscire a fare. Sulla base di questi presupposti, che sono assolutamente necessari a recuperare un minimo di credibilità e freddezza nell'assumere decisioni delicate in una materia come questa, sono allora d'accordo con il presidente Bianco nel procedere ad una sospensione che consenta di potersi misurare sulla decisione del Governo che a me sembra chiarissima, nel senso che la sottosegretario Lucidi ha espresso con chiarezza qual è il senso delle cose che il Governo propone e rispetto a quelle cose noi dovremmo avere il coraggio di misurarci senza infingimenti, consapevoli che siamo portatori solamente di quello che la nostra coscienza ci detta e non di un bagaglio che all'esterno deve essere venduto come maggioranza od opposizione. Rivendichiamo tutti la capacità di una analisi concreta delle cose che dobbiamo decidere e poi, invece, arriviamo in Aula e dobbiamo assistere ad una cristallizzazione che io, su materie come queste, considero assolutamente ingenerosa. La sicurezza, il rispetto delle norme comunitarie per l'integrazione sono patrimoni che appartengono alla maggioranza e all'opposizione, e all'interno di questi patrimoni condivisi dovremmo recuperare la capacità di muoverci. Questo, purtroppo, signor Presidente non è per le cause che io ho indicato. Mi muovo quindi in questa direzione e acconsento, nel senso che esprimo voto favorevole alla sospensione, anche se ritengo che i presupposti iniziali hanno inevitabilmente minato un cammino che non mi sembra assolutamente agevole.

Rispetto a ciò, ho ovviamente bisogno di sentire le valutazioni di tutti i Gruppi.

questo provvedimento. Stanno però accadendo delle cose paradossali. Un Sottosegretario si alza in Aula per rispondere ad un'obiezione del collega Calderoli, che chiedeva come sarà poi applicato il provvedimento, come funzioneranno e se ci saranno ancora o no

stiamo leggendo un'agenzia estremamente preoccupante secondo cui il Ministro della giustizia dichiara che a questo punto è meglio lasciar decadere il decreto. allora un chiarimento dal Governo su come ha intenzione di procedere in questo importantissimo settore, in questa materia che interessa tutto il Paese e non soltanto la maggioranza sfracellata di questo Senato, che forse non c'è più.

che richiamo con serenità. Sono emerse necessità di puntualizzazioni, in particolare una specifica sulla quale sono intervenuti molti senatori;

*(FI)*. Signor Presidente, siamo contrari a questa ulteriore sospensione, perché riteniamo di dover innanzitutto rispettare l'impegno assunto nei confronti della Presidenza e anche del Paese di garantire che nella giornata di oggi il testo Il Governo ha chiesto, qualche ora fa, un approfondimento in Commissione; se vi sono ulteriori esigenze di approfondimento, queste possono essere attivate durante la pausa dei lavori tra le ore 13 e le ore 16, ma riteniamo che dovere istituzionale e dovere politico ci porti a richiamare quest'Aula alla sua funzione, quella di votare. Se poi dietro queste richieste di sospensione

però è evidente che ciò che avviene presso l'opinione pubblica è importante; se mi consente, spesso è ancora più importante di ciò che accade all'interno di quest'Aula. Pertanto, il ministro Mastella credo abbia il dovere di chiarire

che la soluzione più ragionevole al problema del quale pure questo emendamento si fa carico sia rappresentata dall'emendamento 1.300, presentato dal Governo. Si fissa la data certa di ingresso per poi stabilire se sono trascorsi i tre mesi e se può attivarsi la valutazione del prefetto circa la insussistenza delle condizioni del diritto di soggiorno. Quindi, si fissa la data certa di ingresso per stabilire se può essere disposto il provvedimento di allontanamento che ha, come primo presupposto, il fatto che siano trascorsi tre mesi e, come secondo presupposto, l'accertamento che non vi siano le condizioni per l'esercizio del diritto di soggiorno fissate dalla direttiva europea e recepite dal decreto legislativo 6 Pensare, invece, ad un dovere di segnalazione della propria presenza sul territorio nazionale a fini di pubblica sicurezza, scaduti i tre mesi di soggiorno libero, significa introdurre una limitazione alla libertà di movimento e all'esercizio del diritto di soggiorno previsto dalla normativa europea, che è in netto contrasto con lo spirito e con la lettera della direttiva europea,

nel processo di formazione e di rafforzamento delle istituzioni europee, compresa la determinazione dei princìpi della Costituzione europea. Colleghi come Giuliano Amato, Gianfranco Fini e Lamberto Dini sono stati protagonisti di questo processo. Chiedo a tutti i colleghi di mantenersi coerenti e fedeli alle scelte che rappresentano un punto di riferimento cardinale e al di sopra delle parti per la politica estera del nostro Paese. Una scelta fondamentale è stata quella di condividere le direttive europee, il loro impianto, lo spirito che le anima, le norme che da esse derivano. Tra queste norme c'è anche quella che stabilisce le condizioni del diritto di soggiorno: la direttiva europea dà al prefetto un potere discrezionale di valutazione che deve essere volto anche ad accertare se vi sono, il fatto che lo straniero manchi di reddito, condizioni di integrazione per cui si può non ricorrere al provvedimento di allontanamento. In questo quadro, credo che la segnalazione della propria presenza sul territorio nazionale italiano non possa essere prevista, se non come un onere finalizzato all'esercizio del diritto di soggiorno nelle due forme diverse: quella anteriore ai tre mesi di permanenza e quella che si prevede successivamente ai primi tre mesi di permanenza. Pertanto l'emendamento 1.27 non è condivisibile, mentre è preferibile conseguire lo stesso risultato e lo stesso obiettivo, anche in termini di potenziale tutela della sicurezza, attraverso l'emendamento presentato dal Governo. [BOCCIA

in cui uno degli Stati dell'Unione Europea può richiedere ad un cittadino straniero di certificare alcune condizioni della sua permanenza nel territorio di quello Stato, Stato, dalla data del suo arrivo all'iscrizione all'anagrafe o all'accertamento delle sue fonti di sussistenza e delle risorse economiche di cui gode;

ha carattere imperativo cioè non rientra tra quelli della pubblica sicurezza. Ieri il ministro Amato, nell'illustrare la posizione del Governo,

che è impossibile dare a questa certificazione il valore di un atto che ha effetti irremovibili, poiché questo

entro i cardini della civiltà e della cultura del diritto, dei princìpi costituzionali e, soprattutto, di quelle acquisizioni

e volge a rendere certo l'ingresso nel nostro Paese, mentre la dichiarazione anagrafica, che si rende dopo i tre mesi, rischia di non poter essere mai valutata nel termine poiché non esiste alcuno strumento per sapere se questo soggetto comunitario è entrato nel nostro Paese con una data certa.

e che quindi la questione aveva già trovato una sua intesa all'interno della Commissione. Non posso dunque che insistere nei confronti dei colleghi affinché ritirino l'emendamento

l'emendamento, così come proposto, attraverso una propria specifica riformulazione che sostanzialmente sostituisce la parola «redditi» con «fonti», che è ovviamente più propria e corretta.

sicurezza nel Paese. Abbiamo tutti il dovere di capire se le scelte che compiamo di intervento normativo sono coerenti o meno con la direttiva europea; altro può essere - e mi sembra che su questo lo stesso Ministro, ma non solo, anche la disponibilità ad accogliere gli ordini del giorno presentati dall'opposizione lo ha confermato - porre in sede europea la questione che questa direttiva può non essere sufficiente a favorire un sistema in grado di reagire a situazioni problematiche.

di Stato per l'interno*. Grazie, Presidente. Vorrei richiamare all'attenzione dell'Aula una sentenza della Corte europea del 23 marzo 2006 che conferma quello che vi dicevo, cioè che con questo emendamento l'Italia verrebbe sottoposta a procedura d'infrazione. La Corte europea, in regime della precedente normativa

La censura che veniva posta riguardava l'ordine di lasciare il territorio che era stato notificato ad un cittadino per non aver prodotto i documenti richiesti per il rilascio di un titolo di soggiorno entro un dato termine. La Commissione aveva addebitato alla normativa belga il fatto che la mancata produzione da parte del cittadino di uno Stato membro, entro un dato termine, dei documenti giustificativi necessari al rilascio della carta di soggiorno della carta di soggiorno comportasse automaticamente la notifica di un ordine di allontanamento, ritenendo che venisse in tal modo pregiudicata la sostanza stessa del diritto di soggiorno direttamente attribuito dal diritto comunitario. Rispetto a questo si è pronunciata la Corte europea, confermando che la mancata presentazione dei documenti non poteva ritenersi ragione di allontanamento dal territorio. Credo che la direttiva europea lo dica con chiarezza.

conto, signor Presidente,

tra l'altro con un avvio che sapeva di razzismo e di intolleranza, quando abbiamo visto ruspe con telecamere al seguito evidenziare al popolo italiano dov'era il problema della sicurezza e dove si trovavano i colpevoli. In questo caso mi è d'obbligo ricordare (non lo si fa mai, ma credo lo si debba fare) il famoso triangolo marrone. Pochi lo sanno, ma il triangolo marrone

senza attenzione ha voluto lanciare una certa campagna, di cui si è immediatamente pentito, ovviamente, perché quando si scopre un vaso e non si sta sulla razionalità e sulla serietà delle cose,

di una persona della stessa comunità. Veniamo al dunque. Credo che in parte la discussione sia alterata dal non tener conto che comunque le direttive europee, piacciano o non piacciano, non sono fatte per il restringimento. Le norme europee e l'Unione Europea che abbiamo costruito hanno come presupposto il garantire, ripeto, garantire a tutte le popolazioni interne all'Unione Europea la libera possibilità di viaggiare, di visitare e di abitare in qualsiasi Paese che ne faccia

e dalle interviste in televisione. Specie su temi che attengono alla libertà, alla circolazione, alla cultura e alla costruzione di una cittadinanza europea, si deve, secondo me, sempre stare all'interno della rigorosa della rigorosa normativa europea e della costruzione di una cittadinanza che ci deve vedere, comunque non come estranei ma persone gradite sul nostro territorio e che con il nostro territorio costruiscono

votato. Concentriamo l'attenzione sul comma 02, perché su di esso il Ministro dell'interno, ieri, e il Sottosegretario per l'interno, oggi, pongono questioni che meritano attenzione da parte di tutta l'Aula. Il Ministro e il Sottosegretario dicono comma 02 si pone in contrasto con la direttiva n. 38 del 2004 e che addirittura esso fa rischiare una procedura di infrazione. Mi permetto anzitutto di dire, Presidente,

decidono di assumere un atteggiamento leale nei confronti dello Stato ospitante, iscrivendosi all'anagrafe e pagando i contributi, perché vi è l'esigenza di non gravare sui bilanci dello Stato ospitante e così via.

non si dichiara, non ha nessuna intenzione di farlo, vive ai margini e così facendo viene attratto o dall'area dello sfruttamento in nero o addirittura dall'area della clandestinità. Un'ipotesi del genere è così conforme alla direttiva che l'articolo 9, comma 2, del decreto di recepimento la prevede esplicitamente. Noi ci limitiamo con questo a qualificare il comportamento di coloro che non adempiono a questo dovere di lealtà fondamentale nei confronti dello Stato ospitante dello Stato ospitante come lesivo della sicurezza pubblica. Cosa c'è di scandaloso e antieuropeo in tutto questo? Se ciascuno di noi, abbia o non abbia l'immunità parlamentare, va in una stanza di albergo è obbligatoria o no la dichiarazione in questura della sua presenza? E siamo cittadini italiani.

per il comunitario che non intende ottemperare a quest'obbligo di fondamentale lealtà? A proposito poi dell'infrazione, onorevole Lucidi, la sua citazione di una sentenza della Corte di giustizia, come direbbe un Ministro di questo Governo, non ci azzecca nulla, perché questa fa riferimento all'articolo 5, comma 4, della direttiva, cioè all'obbligo di presentare i documenti di colui che si è dichiarato, qui stiamo prendendo in considerazione il comportamento di chi non si dichiara, di chi non si fa riconoscere, della persona della cui identità nessuno sa nulla. Ma allora come non ritenere la violazione di un obbligo di questo tipo lesiva dei motivi di pubblica sicurezza? Mi rendo conto, signor Presidente, che questo è un passo ulteriore rispetto al decreto di recepimento della direttiva, ma ci vuole coraggio a dire che è contro di essa: è certamente conforme allo spirito della direttiva.

e cioè che non fissa nessuna sanzione rispetto all'inottemperanza dell'obbligo di dichiarare la presenza, e noi sappiamo che il precetto senza sanzione può essere un garbato invito, un'omelia, una predica, ma non è nulla di giuridicamente vincolante. In conclusione, signor Presidente, per tutte queste ragioni, io credo che ci sia motivo da parte di tutta l'Aula per votare un emendamento che in alcune parti ha ricevuto il consenso del Governo (tant'è vero che ne ha fatto fotocopia in un proprio emendamento) per altro verso, è assolutamente conforme alle norme di quell'Europa che non tollera che al proprio interno ci siano l'impunità e la violazione delle regole, ma che esige il rispetto di quel dovere fondamentale che consiste nel dichiararsi nei confronti di chi ospita.

l'emendamento 1.300 rappresenta un confine oltre il quale la sua azione, l'azione del Governo, non può e non ha la possibilità di andare. Infatti, egli ha sottolineato come quella dell'emendamento 1.300 non possa risultare come dichiarazione con finalità di sicurezza e di ordine pubblico,

tende oggettivamente a tenere distinto il canale dell'espulsione per ragioni di sicurezza da quello dell'allontanamento per violazione degli obblighi legati alla pura presenza sul territorio.

1.27 (testo 2) esistano in termini oggettivi una serie di punti di riferimento che per certi versi possono essere condivisibili,

quanto riguarda la definizione e la modifica della normativa e della direttiva europea, che rappresentano secondo noi il vero limite della nostra discussione e riflessione.

sul complesso degli emendamenti e sul senso di quello che si vuole perseguire da parte dei colleghi dell'opposizione. Noi stiamo discutendo molto, in questa sede, della conformità alla direttiva europea, ed è certamente questo un punto colto con esattezza, perché è il parametro principale, insieme ovviamente ai profili della costituzionalità per il diritto interno. Lo è, tuttavia, in un senso che va colto a pieno

Il problema non è se si possa attivare o meno la procedura d'infrazione, che è certamente possibile: la questione veramente in gioco riguarda, piuttosto, un profilo ben più pregnante di certezza del diritto. Perché è assolutamente decisivo tenere in debito conto la conformità alla direttiva e, in particolare, a questa direttiva? Perché questa è una direttiva, come si dice in gergo, *self-executing*, cioè di diretta applicazione. Come i colleghi sanno,

Ma alcune direttive, soprattutto nella fase più recente dell'esperienza dell'Unione Europea, sono autoapplicative per la specificità delle proprie prescrizioni:

arrivare poi, nel momento dell'applicazione, anche alla prospettiva non già dell'impugnativa in sede europea, ma a quella della disapplicazione da parte del giudice nazionale. infatti, di un contesto nel quale il giudice nazionale procede direttamente all'applicazione del diritto europeo e quando la norma di diritto interno

di elevata incertezza del diritto, perché conduce alla diretta disapplicazione della norma interna che non sia conforme alla direttiva. Essendo questo un tipico contesto

l'omogeneità va riferita al cittadino comunitario che entra e al cittadino nello Stato nazionale. Questo è il termine corretto del paragone. Pertanto, se c'è una

ci troviamo in una condizione antigiuridica che, non solo conduce all'infrazione, ma anche alla possibile disapplicazione della normativa nazionale.

risulterebbe precluso o addirittura assorbito l'emendamento 1.302 del Governo, perché la sua formulazione sarebbe assolutamente identica.

chiedo scusa ai colleghi se rischio di essere pedante. Mi dispiaccio per la loro intolleranza, ma credo di affrontare una questione assai seria, che dal punto di vista procedurale rischia di portare ad effetti che noi abbiamo il dovere di

noi. Pongo la questione della chiarezza anche come un problema di regole di comportamento all'interno dell'Aula. Pretendo la chiarezza per evitare una discussione e una lite, ma questo richiede buonsenso e non un atteggiamento di inutile intolleranza, che produce soltanto guai e rischia di portarci

senatore Salvi

il nostro emendamento votando per parti separate l'emendamento 1.27 riferito alle fonti certe, lecite e così via, non vuole essere qualcosa di sostitutivo a quanto proposto dal Governo. E' il Governo che ha presentato qualcosa

Prego

hanno giustamente evidenziato nei loro interventi, stiamo discutendo un provvedimento di enorme rilievo, perché riguarda la presenza di cittadini comunitari nel nostro Paese nei confronti dei quali quali ci accingiamo a varare norme che possono prevedere misure restrittive della loro libertà personale.

francese, tedesco, britannico o spagnolo (prendo in considerazione questi tre grandi Paesi europei, che per storia, affinità politiche, culturali e democratiche possono essere considerati più vicini alla cultura, alla civiltà, al senso del diritto del nostro Paese) norme non analoghe, ma identiche, che possono riguardare cittadini italiani che vanno

un nostro figlio o una nostra figlia che vivono a Londra o a Parigi di lavori saltuari siano in grado di dimostrare, se fermati dalle autorità di polizia britanniche o francesi, o francesi, le fonti certe del loro reddito, della loro sussistenza, e se sia giusto che un cittadino italiano che si trovi in territorio francese, britannico, spagnolo o tedesco possa essere sottoposto alle stesse misure di restrizione delle libertà personali a cui noi sottoponiamo un cittadino comunitario nel nostro Paese. Io penso (lo dico sulla base della mia grossolana conoscenza del diritto civile e penale di quei Paesi) che ciò non avvenga, però vorrei avere una risposta compiuta da parte del Governo. La domanda posta dal senatore Angius ha certamente un fondamento. Naturalmente, questi problemi sorgono quando si decide di fare un decreto-legge entro un'ora perché è stato commesso un grave crimine e qualcuno lo chiede. Se invece ci si pensa prima, tutti questi problemi vengono esaminati in modo più sereno e disteso e non c'è bisogno di affrontare convulsi dibattiti.

Si sta votando sul testo che è stato distribuito?

si è iscritta all'università francese di Aix-en-Provence, facoltà di diritto internazionale. Tra i documenti che questa ragazza ha dovuto produrre al sindaco di Aix-en-Provence vi sono: la busta paga originale del padre,

dell'appartamento dove questa ragazza doveva andare a vivere; il contratto stipulato con la società elettrica. Senza quei documenti, la ragazza non avrebbe avuto il permesso di restare ad Aix-en-Provence per studio, ma avrebbe avuto semplicemente il visto trimestrale per turismo e vi assicuro che suoi amici italiani qualche mese più dopo aver divelto alcune panchine in un parco pubblico francese, sono entrati direttamente e sono rimasti per sette mesi nelle patrie galere francesi. Ora, vi dico che sono certo che questa ragazza mi abbia raccontato la verità, perché è mia figlia e ho dovuto portare al sindaco di Aix-en-Provence la busta paga della Camera dei deputati, perché non gli importava niente che suo padre fosse un deputato: voleva la prova che quella ragazza avesse i soldi per mantenersi.

esprimo semplicemente il mio dissenso rispetto al voto che la maggioranza si accinge ad esprimere, nel senso che sono contrario e sarò contrario a tutte le norme, anche successive, che introducono nell'ordinamento italiano, e solo nell'ordinamento italiano, misure che costituiscono limitazioni delle libertà che non esistono in altri Paesi.

questo punto: dopo le parole «risorse economiche sufficienti» inserire le altre «derivanti da fonti lecite e dimostrabili». Votiamo soltanto questo? Chiariamo,

A me pare però che in quell'espressione vaga «derivanti da fonti lecite dimostrabili» possa individuarsi un'inversione dell'onere della prova. Comunque, non vi è chiarezza sul testo. Qualunque giurista sa che sarebbe bene precisare i testi, ma

Presidente, mi verrebbe da dire che chiedo la parola sul disordine dei lavori, perché è destino di questa seduta che colleghi, dell'uno e dell'altro schieramento, rivolgano richieste di chiarimenti al Governo e il Governo non risponda. Non voglio sostituire il Governo, ma solo far notare che l'articolo 7 della direttiva europea n. 38 del 2004 e l'articolo 7 del decreto di recepimento indicano come condizione precisa, per la presenza nel territorio nazionale oltre i tre mesi, il disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti.

di produrre la documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i familiari. Risorse evidentemente lecite. Quindi... RUSSO

Evidentemente lecite, perché sarebbe davvero singolare che in una direttiva si scrivesse «risorse economiche sufficienti lecite o illecite che siano».